La seduta è aperta

Dichiaro aperta la votazione.

L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Senatrici e senatori, è deceduto nella tarda serata di ieri a Roma, all'età di 93 anni, il senatore a vita Emilio Colombo, protagonista della vita politica italiana del dopoguerra e componente autorevole di questa Assemblea. Deputato all'Assemblea Costituente, esponente di spicco della Democrazia Cristiana, Emilio Colombo è stato Presidente del Consiglio, più volte Ministro e Presidente del Parlamento europeo. Nominato senatore a vita nel 2003 dal presidente Ciampi, il senatore Colombo è stato Presidente provvisorio dell'Assemblea del Senato nelle prime due sedute di questa nostra legislatura. La sua figura sarà solennemente commemorata dal Senato in un'apposita e prossima seduta. Avremmo dovuto presentare prossimamente in sala Zuccari il suo libro «Per l'Italia, per l'Europa». lo faremo senza di lui, ma in ricordo della sua straordinaria figura. Nel manifestare il cordoglio della Presidenza e di tutto il Senato, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento.

approfondita e complessiva del quadro generale, con una visione delle opere infrastrutturali che servono all'Italia. Non è pensabile, infatti, né immaginabile lo sviluppo del nostro Paese fuori da interconnessioni con reti e corridoi che devono sostenere, con logistiche adeguate, gli imponenti flussi di traffico persone, merci e servizi e, insieme a questi, anche le economie e la coesione territoriale e sociale nel nostro Paese, tra gli Stati europei e con i sistemi di altri Paesi confinanti. Per quanto riguarda le scelte di fondo, come ha avuto anche modo di assicurare il ministro Lupi in sede di Commissione, nessuna Regione italiana può rimanere e resterà indietro. In particolare, il tema della cooperazione tra le Regioni adriatiche è posto all'attenzione ministeriale e di Governo sin dagli anni Novanta, quando fu costituita l'Iniziativa Adriatico Ionica tra l'Italia e i Paesi dei Balcani occidentali. Con questo nuovo approccio macroregionale, sviluppato soprattutto nel corso degli ultimi anni, la cooperazione economica e culturale ha acquistato un notevole rilievo, grazie soprattutto all'impegno delle Regioni adriatiche italiane, che hanno creduto e scommesso sulle opportunità offerte dalla mutata realtà geopolitica dei Balcani occidentali già alla fine degli anni Novanta. In questa prospettiva, i progetti di cooperazione territoriale, sostenuti anche dalla politica di coesione europea, rappresentano un'opportunità imperdibile per recuperare le differenze e gli squilibri ancora esistenti e per accompagnare la politica di ripresa economica e di crescita dell'occupazione. La prossima programmazione finanziaria 2014-2020 a livello europeo apre quindi un nuovo capitolo strategico nella cooperazione territoriale e rappresenta un'opportunità che il Governo intende ovviamente cogliere appieno e prontamente.

l'Europa, assume la dimensione finanziaria di 29,2 miliardi di euro. Tale somma è così ripartita: per quanto riguarda i trasporti 23,1 miliardi

della dotazione finanziaria del meccanismo per collegare l'Europa, con rischi anche relativamente alla possibilità del finanziamento nella misura massima prevista dal regolamento, riteniamo ci siano ancora tutte le condizioni per realizzare una rete prioritaria che rispetti gli ambiziosi requisiti indicati nelle linee guida e nella programmazione. Per questo, nell'ambito del processo di codecisione sui nuovi regolamenti relativi alle reti TEN-T, il Ministero per le infrastrutture e per i trasporti si è fatto promotore di numerose iniziative per sostenere l'estensione del corridoio Baltico-Adriatico verso Sud, l'inclusione della linea ferroviaria adriatica nella rete centrale (la rete *core*), per il suo significato di raccordo del sistema portuale e di complementarità nei flussi di trasporto merci tra Nord e Sud lungo la dorsale adriatica. Sono già stati ottenuti parziali successi. Infatti, allo stato attuale, la sezione compresa tra Trieste e Ravenna, in quanto parte del corridoio Baltico-Adriatico, appartiene alle rete centrale, così come la sezione ferroviaria Bologna-Ancona, che fa parte del corridoio Helsinki-La Valletta, e la sezione Napoli-Bari-Taranto. Per contro, la sezione a sud di Ancona, fino a Foggia, risulta compresa nella rete TEN-T *comprehensive*, cioè nella rete globale, così come la sezione da Bari fino a Lecce. Il tema dell'inclusione dell'intero tracciato della linea costiera adriatica è stato affrontato in numerose occasioni, a partire dall'incontro bilaterale tenutosi a Bruxelles il 6 maggio 2011. Successivamente, la richiesta è stata riproposta nelle riunioni del Consiglio europeo del 19 aprile, del 4 maggio e del 7 giugno 2012. L'esito del negoziato non ha consentito, finora, di ottenere per intero l'inserimento della linea ferrovia adriatica nella rete centrale in quanto la rigorosa metodologia europea non consente la connessione di nodi prioritari all'interno della rete centrale mediante rami di rete che presentino tracciati paralleli tra di loro, come avviene, nel caso di specie, tra la dorsale centrale alta velocità/alta capacità e la linea adriatica. L'inclusione della linea adriatica nella rete centrale

al corridoio prioritario Helsinki-La Valletta e quindi alla rete *core*, mentre la sezione Bari-Lecce in quanto connessione di un nodo *core*, quello di Bari, con un nodo non avente le caratteristiche di nodo prioritario, Lecce, non è includibile nella rete centrale e, conseguentemente, in un corridoio prioritario. In conclusione, rispetto all'intero tracciato della linea Milano-Lecce, le sezioni comprese tra Ancona e Foggia e tra Bari e Lecce risultano, ad oggi, incluse nella rete TEN‑T *comprehensive*, la rete globale, e pertanto possono concorrere all'ottenimento di contributi comunitari, sia pure nella misura del 5 per cento dei fondi disponibili, nonché all'utilizzo degli strumenti innovativi finanziari quali i *project bond* previsti nella prossima programmazione. Una strategia di crescita dei distretti produttivi consente infatti una maggiore articolazione fra i diversi strumenti di intervento a disposizione dell'Unione europea, al di là dei meri stanziamenti destinati alla politica di coesione. Questo vale, in particolare, per la Banca europea per gli investimenti che, con le dovute garanzie, si può anche aprire a realtà regionali e soprattutto a realtà macroregionali. la dorsale adriatica non risulti per intero nella rete TEN-T *core*, si può affermare che i porti italiani prioritari che si affacciano sulla costa adriatica sono raccordati ai predetti corridoi, e precisamente Trieste-Venezia-Ravenna, Il nostro impegno è di promuovere l'inserimento dei centri urbani dei porti adriatici nazionali all'interno di questo corridoio, utilizzando le opportunità offerte dai nuovi regolamenti TEN-T in corso di approvazione che lasciano aperta la possibilità di effettuare periodiche revisioni ‑ la prima, al momento, è fissata al 2023 - delle reti di trasporto di rilievo Esistono quindi le premesse affinché la programmazione europea del prossimo programma quadro assicuri il sostegno finanziario agli investimenti che saranno ritenuti compatibili con l'attuale situazione di bilancio e che siano volti a dare attuazione alle potenzialità espresse dal sistema portuale e interportuale Adriatico-Ionico, che svolge un ruolo strategico, importante per l'approvvigionamento e l'accesso ai mercati esteri non solo delle regioni che affacciano al mare Adriatico ma di tutto il Mediterraneo e del Medio Oriente. Ovviamente noi ci impegniamo ad un tavolo tra Ministeri, Regioni e Ferrovie per cercare di portare a casa il miglior risultato possibile.

delicati, così vasti e problematici, che vanno inseriti in un dibattito più articolato e ampio, che riguardi

ogni iniziativa in sede europea per promuovere il prolungamento del corridoio baltico-adriatico (n. 1) lungo la direttrice Ancona-Pescara-Bari-Taranto-Lecce, che costituisce un elemento strategico strategico tra i diversi poli produttivi e le aree portuali dell'Adriatico, capace di rendere l'Italia il baricentro dei traffici commerciali tra l'Oriente e l'Occidente, nonché fra i Paesi del Nord Europa e le nuove economie che si affacciano sul Mediterraneo», il parere del Governo è favorevole. Per quanto riguarda

in favore di progetti indirizzati all'ammodernamento della linea ferroviaria della dorsale adriatica, con particolare riferimento alla direttrice Milano-Lecce, in considerazione della della programmazione delle risorse dell'UE per il periodo 2014-2020», le seguenti: «nel quadro dei fondi comunitari che verranno messi a disposizione per le politiche di trasporto»,

il parere è favorevole con la seguente riformulazione: «impegna il Governo ed in particolare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a verificare le condizioni per la realizzazione di opere prioritarie di adeguamento e velocizzazione della linea ferroviaria Pescara-Roma».

Signora Presidente, prendiamo atto della volontà espressa dal Governo di ridiscutere in sede più ampia e completa il problema da noi posto.

l'8a Commissione: «L'obiettivo che intendo perseguire è quello di evitare che nel Paese ci siano servizi di serie A e di serie B, ci siano, ancora peggio, aree territoriali di serie A e di serie B». a pagina 44 afferma: «Il "diritto alla mobilità", previsto all'articolo 16 della Costituzione, rappresenta un obiettivo chiave del Governo». Noi speriamo che la volontà espressa oggi dal Governo e quanto scritto dal Ministro in questo testo siano consequenziali e che, a breve, si possa aprire un dibattito serio e compiuto per decidere una buona volta cosa vuol fare l'Italia di questa parte del

Presidente, senatrici e senatori il ritiro della mozione a prima firma del senatore Compagnone mi facilita nel compito di dare un giudizio estremamente tranciante tranciante rispetto alle proposte che essa conteneva. Ovviamente anche il pronunciamento elettorale delle popolazioni direttamente interessate a quella sciagurata proposta del ponte sullo Stretto di Messina nei giorni e nelle ore scorsi ha risposto in maniera

risente di un'impostazione che ha il riferimento nel Moloch delle grandi opere.

su un quadro strategico della rete innanzitutto ferroviaria e poi di tutto il sistema Italia all'interno del sistema Europa, che tenga conto della dimensione della macroregione adriatico-ionica, con le interconnessioni e il diritto alla mobilità lungo tutta la dorsale, anche in termini di

fare qualcosa significa comprometterne un'altra. Fare un investimento forte sul ferro e sul trasporto locale significa

nella consapevolezza della straordinaria importanza di un'efficace rete logistica ed infrastrutturale di collegamento tra regioni remote d'Europa che favorisca la mobilità di persone e merci e il conseguente indotto,

è allo stato difficilmente realizzabile. Anzi, in un momento socio‑economico come quello che stiamo attraversando direi che è quasi impossibile, difficilissima è quasi inutile pensarle certe cose. ma soprattutto da cittadino e osservatore obiettivo della realtà economica attuale, non posso non sottolineare quanto possa rivelarsi sbagliato mettere in cantiere, con l'incertezza e l'approssimazione che deriva da una mozione, da ordini del giorno o da documenti come quelli alla nostra attenzione questa mattina, altre opere come quella sulla quale ci apprestiamo ad esprimerci: una mozione, un ordine del giorno,

quanto possa ciò essere odioso in un momento in cui è già difficile reperire risorse per portare a termine le infrastrutture già cantierate, già in fase di realizzazione e in attesa di finanziamento e che tanto fanno

Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'Adriatico è un mare semichiuso e i Paesi che vi si affacciano hanno una comune radice storica e una omogenea cultura. il «mare dell'intimità», come lo definisce lo scrittore croato Predrag Matvejević, secondo il quale «nei tempi più antichi coloro che approdavano sulle sue sponde si trovavano in imbarazzo: è un golfo o un mare?» Queste caratteristiche non possono non agevolare le politiche di sviluppo regionale promosse dall'Unione europea. Le macroregioni europee sono ormai una realtà: mi riferisco alla macroregione baltica, a quella danubiana e, appunto, a quella adriatico-ionica. A dicembre, infatti, il Consiglio europeo ha dato formalmente mandato alla Commissione europea di avviare la strategia operativa che nel 2014 porterà alla creazione della suddetta macroregione. La nomina, poi, del presidente della Regione Marche alla guida dell'Intergruppo adriatico-ionico del Comitato delle Regioni d'Europa è un elemento significativo nel percorso di delineazione della *road* *map* che ne porterà alla costituzione. Del resto, negli ultimi tempi l'Iniziativa adriatico-ionica schema di cooperazione regionale che abbraccia otto paesi (Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia, Serbia, Albania, Montenegro e Grecia), tenuto a battesimo nel 2000 con la Carta di Ancona e con sede operativa nel capoluogo regionale, ha infatti accelerato la marcia che porta alla macroregione. Dieci anni dopo, il quadro geopolitico in cui opera l'Iniziativa adriatico-ionica è profondamente mutato; tuttavia le ragioni che hanno determinato l'istituzione della IAI hanno mantenuto se non accresciuto la loro validità nel corso degli anni. L'accoglienza dei Paesi balcanici e della Turchia nella famiglia europea è una sfida da cogliere e vincere, se l'Unione vuole veramente svolgere un ruolo di più alto profilo nel mondo, se si mira ad esercitare una maggiore influenza nel Caucaso, in Asia centrale, in Medio Oriente e nel Mediterraneo se si vuole recuperare competitività economica e garantire sicurezza energetica. Per realizzare ciò, abbiamo bisogno quindi di una strategia europea per l'Adriatico e lo Ionio, e lo Ionio, che comprenda tutti i Paesi della regione e ciò in sintonia con l'approccio dell'Unione europea alle macroregioni, filosofia con cui l'Italia è pienamente d'accordo. In tal senso voglio ricordare la recente posizione assunta, lo scorso 27 maggio, dal vice ministro degli affari esteri Marta Dassù, a Bruxelles, nel corso della quindicesima riunione dei Ministri degli affari esteri dell'Iniziativa adriatico-ionica: ella ha individuato come priorità dell'Italia, in vista del suo semestre di presidenza della Unione europea nella seconda metà del 2014, la realizzazione del Piano d'azione per la strategia adriatico-ionica quale strumento per rafforzare la coesione europea in un'area cruciale per la stabilità dell'intero continente. che tutto ciò sia accompagnato, per evitare che il progetto nasca monco, da un recupero nel campo delle infrastrutture materiali che debba comprendere tutti i settori: viario, ferroviario e marittimo. Il Governo, come si chiede in questa mozione, deve porre in essere tutte le iniziative necessarie affinché si preveda una prosecuzione del percorso dell'alta velocità nel corridoio 1, oggi fermo ad Ancona (secondo l'emendamento votato nel dicembre scorso dalla Commissione trasporti del Parlamento europeo e in attesa della ratifica con il voto finale dello stesso), lungo la dorsale adriatico-ionica fino a giungere a Lecce. Il prolungamento del corridoio 1 potrebbe aprire nuovi scenari anche per i distretti economici presenti lungo l'Adriatico, favorendo l'*import* e l'*export* in una porzione di Europa più ampia che sembra risentire meno della crisi economica in atto, con un sistema produttivo in fase espansiva, facendo del Mediterraneo e dell'Italia una grande piattaforma logistica e il baricentro dei traffici commerciali tra l'Oriente e l'Occidente. Il potenziamento e rafforzamento della mobilità su ferro assume quindi una duplice veste: da una parte consentirà un servizio finalmente adeguato per quel che riguarda il trasporto dei passeggeri; dall'altra, una mobilità molto più veloce per il trasporto merci. Si aumenterebbe quindi la coesione territoriale in termini di crescita e competitività. Attraverso l'indispensabile adeguamento dell'infrastruttura ferroviaria lungo la direttrice Milano-Lecce si favorirà anche il rilancio di una zona ad alto potenziale economico sia per quanto riguarda diversi poli produttivi che per le aree portuali dell'Adriatico. Attualmente la distribuzione dei traffici in questa zona è nettamente sbilanciata a favore del trasporto su strada; la realizzazione del corridoio potrebbe avere come primo effetto quello del riequilibrio dei flussi di traffico portando una maggiore quota di merci verso la ferrovia, modalità più amica dell'ambiente rispetto alla strada. Come detto, l'asse ferroviario in oggetto non costituisce però un'importante infrastruttura solo per le merci, ma dalla sua implementazione può trarre enorme vantaggio anche il trasporto dei passeggeri. Lungo il tracciato del corridoio Baltico-Adriatico si trovano, infatti, numerosi agglomerati urbani e ciò potrebbe influire anche per il miglioramento dei flussi turistici per tutte le Regioni interessate dal corridoio 1. È giunto È giunto il momento di cambiare culturalmente il modo di fare trasporti: bisogna investire di più sul ferro, non solo perché è il mezzo più ecosostenibile, ma anche per evitare la saturazione delle strade. Nell'immediato bisogna investire per aumentare l'efficienza; nel medio e lungo periodo occorre iniziare

preveda il prolungamento di quello Adriatico-Baltico fino al Sud. In secondo luogo, serve immaginare un progetto nazionale coordinato con i progetti dell'Europa, impegnandosi poi affinché si ottenga da questa il suo pieno riconoscimento e sostegno. Il meccanismo per collegare l'Europa prevede un investimento di 31,7 miliardi di euro per ammodernare le infrastrutture di trasporto europee, costruire i collegamenti mancanti ed eliminare le strozzature. Ciò comprende 10 miliardi di euro accantonati nel Fondo di coesione per progetti di trasporto nei Paesi della coesione, mentre i rimanenti 21,7 miliardi sono stati messi a disposizione di tutti gli Stati membri per investimenti nelle infrastrutture di trasporto. Altresì, bisogna però considerare come prioritarie alcune opere per il potenziamento degli assi viari; mi riferisco in modo particolare a due direttrici fondamentali: Livorno-Ancona, con l'importante infrastruttura Fano-Grosseto, e Ancona-Roma. Per quel che riguarda la prima opera, Toscana, Umbria e Marche hanno firmato un'intesa per la costituzione di una società pubblico-privata che la realizzi utilizzando l'innovativa modalità del contratto di disponibilità. Anche la Banca europea per gli investimenti contribuirebbe al progetto e il Ministero delle infrastrutture si è già detto disponibile a considerarla opera d'interesse nazionale. In conclusione, signor Sottosegretario, l'adeguamento e il potenziamento delle infrastrutture materiali, siano esse viarie, ferroviarie o portuali, comporterebbero notevoli benefici in termini di servizi alla persona, al tessuto imprenditoriale esistente, alla capacità di attrazione di flussi turistici e potenziali nuove attività economiche e un innegabile salto di qualità per permettere a molte delle nostre Regioni, all'interno del progetto della macroregione adriatico-ionica, di costruire un ponte fra i Paesi del mar Mediterraneo e il Nord-Europa. Infine, signor Sottosegretario, un ricordo particolare: vengo da Matera, una città che non è assolutamente bagnata dal mare (e non vorrei che questo fosse un difetto) e che continua ad essere l'ultimo capoluogo di provincia non ancora raggiunto dalle Ferrovie dello Stato.

che interviene sulla necessità di un'adeguata infrastrutturazione della dorsale adriatica, il punto per noi controverso è quello in cui si chiede il prolungamento del corridoio Baltico-Adriatico in un contesto in cui le attuali reti di collegamento ferroviario sono a tratti fatiscenti e a tratti addirittura inesistenti. Il nostro dubbio è e resta come si possano programmare opere straordinarie di miglioramento in assenza di una condizione di base essenziale e necessaria. Per i motivi sopra detti la nostra intenzione di voto riguardo tale

bene il testo della mozione e ne vogliamo parlare anche alla presenza del Sottosegretario, visto che ritiene la tematica così importante da meritare una discussione più ampia. Innanzitutto, non riusciamo a capire

totalmente in secondo piano gli argomenti introduttivi sui corridoi europei (questa sì che è una tematica di maggiore importanza). Da parte nostra è impossibile non seguire un'uniformità di pensiero riguardo al tema che abbiamo da sempre sostenuto con tutte le nostre forze: una ferma e decisa opposizione alla realizzazione del ponte di Messina, e non per capriccio o per partito preso,

come sintetizzato dai grafici dell'Istituto nazionale di geofisica. La cantierizzazione dei cospicui tratti costieri comporterebbe l'alterazione di *habitat* marini unici nel Mediterraneo, andando ad alterare la flora dei medesimi ambienti; si tratta di un'area ampiamente vincolata per gli straordinari valori paesaggistici e severamente tutelata dall'Unione europea.

per arrivare poi nella mia Sicilia dove le infrastrutture primarie ancora oggi non esistono, dove non esiste un minimo di sistema di infrastrutture che possa legare bellezze architettoniche, culturali e ambientali fondamentali per la crescita e lo sviluppo di quei territori. Ve ne cito solo alcuni: Segesta, Selinunte, Agrigento, Taormina, l'Etna, le Egadi e le

ma alcuni di voi, qua dentro, hanno delle responsabilità: qualcuno di voi era già qua dentro quando quelle decisioni sono state prese - mi piacerebbe cominciare a capirlo, facendo nomi e cognomi, chi sono i responsabili di così tanto sperpero di denaro pubblico.

si parlava di lavoro e la collega si emozionò per quell'intervento. La mancanza di sensibilità sta appunto in questo: cerchiamo di spiegare bene perché giovedì scorso non si è deciso di votare queste mozioni così diverse; cerchiamo di capire perché il «modello unico», tutto compatto, ha deciso di spostare questa discussione ad oggi perché era chiaro che due mozioni così differenti non potevano essere unite. Probabilmente il Gruppo Grandi stava facendo, signori miei, a costo e spese dei cittadini, propaganda elettorale; stava facendo questo, perché domenica si sono

Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, è vero: il dibattito d'Aula serve, scarsamente partecipato, scarsamente frequentato e scarsamente ascoltato. Se infatti il dibattito d'Aula raggiungesse l'obiettivo che si prefigge (ossia promuovere un fecondo rapporto tra differenti posizioni), si costruirebbe o si concorrerebbe a costruire la democrazia. democrazia. Credo che il dibattito fecondo e produttivo, partito da posizioni differenti, che si è sviluppato in merito a questo provvedimento nell'Aula del Senato

perché ho trovato interessante il suo intervento, meno interessante la *vis* polemica in ordine ad un provvedimento su cui non possiamo che dire grazie di un gesto di maturità e di consapevolezza: un gesto di responsabilità a sostegno di un momento importante per la costruzione di un'Italia unita che si presenti più forte nello scenario europeo. Entro un po' nel merito, amici. Il dibattito è stato proficuo, e voglio ricordare la partecipazione del Gruppo PdL alla stesura di questa mozione,

sapendo che ci sono momenti nei quali i principi della divisività non fanno bene alla bandiera tricolore e allo sviluppo di un percorso unitario che ci presenti forti in Europa. Abbiamo quindi partecipato con convinzione alla stesura e all'*iter* di questa mozione, le cui conclusioni oggi condividiamo, perché in momenti come questo la politica è chiamata a trasformare le contrapposizioni e la contesa in un confronto costruttivo, per il bene della collettività. Siamo in piena Siamo in piena fase di confronto a livello europeo, confronto che, nell'ambito della più ampia Strategia Europa 2020, è tutto proteso a disegnare il futuro della politica di coesione ed il suo ruolo essenziale nel contribuire ad una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, promuovendo al tempo stesso uno sviluppo armonioso dell'Unione e delle sue regioni grazie ad una riduzione delle disparità L'Italia deve e può dare un contributo rilevante nell'orientare in maniera sostanziale tale confronto, perché crei le condizioni per rendere più efficace la politica di coesione e per promuovere gli interventi necessari, sul piano dei contenuti e delle regole della programmazione e di attuazione, per conseguire risultati concreti. Caro collega Davico, c'è una cassaforte, il Governo ha ripetuto più volte, e ringrazio per questo il Governo e ancora oggi il Sottosegretario. È una cassaforte aperta, dove ci sono cospicue risorse, che ammontano a oltre 50 miliardi di euro, di cui 29 solo per le infrastrutture: dipende da noi, se vogliamo cogliere questa opportunità o vogliamo dividerci e attardarci su questioni di carattere più generale, talvolta magari scivolando in una polemica inconcludente, e perdere quello che oggi sarebbe utile per il nostro Paese. Non è un caso se oggi siamo qui a discutere una mozione che intende impegnare il Governo sul fronte della promozione in sede europea del prolungamento del corridoio da Lecce ad Ancona, il cosiddetto Baltico-Adriatico, in prospettiva della approvazione della macroregione adriatico-ionica, e su quello della modernizzazione della rete ferroviaria della dorsale adriatica, con particolare riferimento alla direttrice Milano-Lecce, storicamente, atavicamente e assolutamente carente di una adeguata infrastrutturazione che supporti la linea ad alta velocità. Presidente, amici del Governo, spesso in quest'Aula, soprattutto nei momenti importanti, ho la sensazione che si rischi di fare demagogia, quello che non stiamo facendo oggi. «Se non cresce il Sud, non cresce il Paese». Sono dichiarazioni di principio che riscuotono consensi unanimi, ma di fatto poi tardano provvedimenti che siano conseguenti a queste sacrosante dichiarazioni. È una verità che, se non viene sostanziata da interventi concreti nella soluzione del *gap* infrastrutturale, assolutamente insostenibile, rischia di diventare solo un enunziato, demagogicamente esposto, anche con enfasi, per nascondere il perdurante stato stato di egoismo territoriale. Non bisogna dunque perdersi, nella convinzione che si tratti di mero rivendicazionismo. Trovare una soluzione a questo *gap* significa individuare gli interventi, restituendo alla politica di coesione territoriale l'obiettivo che le è proprio, e cioè la promozione dello sviluppo e dunque l'impatto che questi interventi devono poter avere sulla crescita ed il miglioramento della qualità della vita dei territori interessati. L'obiettivo, colleghi, non è il risarcimento di ciò che al Sud è stato levato e che probabilmente neanche le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia hanno riconsegnato a una dimensione autentica di verità; l'obiettivo è quello, peraltro anche evocato dall'articolo 16 della Costituzione, del diritto alla mobilità che deve avere livelli di uniformità sull'intero territorio nazionale, se crediamo ancora in un'Italia una e indivisibile,

di Trenitalia per sostenere di più e meglio le politiche di mobilità all'interno del territorio nazionale con riferimento specifico al Mezzogiorno d'Italia. Trenitalia deve evidentemente agevolare e non ostacolare il diritto del Mezzogiorno a riprendere in mano il filo del proprio destino, reinserendosi nelle rotte dello sviluppo e godendo di pari opportunità rispetto al resto del Paese. Questa prospettiva al Sud, che è prospettiva per l'intero Paese, è preclusa se il bisturi del medico viene affondato non già per intervenire sulla malattia ma per devastare ed accelerare la fine e il perdurante stato di subordinazione economica, sociale e culturale di questa area del Paese. L'ultimo atto si è consumato qualche settimana fa con l'entrata in vigore nel nuovo orario estivo di Trenitalia, che ha ritenuto di non inserire diverse Regioni del Mezzogiorno, come la Puglia, tra le aree idonee ai collegamenti dell'alta velocità ovvero ai collegamenti con i treni superveloci Frecciargento e Frecciarossa. In questa direzione bisogna muoversi e essere conseguenti.

cittadini e imprese di serie B. Come può il Sud entrare nel circuito virtuoso della competitività se non si dota di tutti gli strumenti necessari a consentire a questa area di diventare di diventare zona di attrazione per investimenti e lo sviluppo? Si pensi al turismo *in primis*.

per sostenere quel processo di crescita e sviluppo che tutti auspichiamo e che per l'Italia, anche per i motivi anzidetti, sono necessari per sostenere un'Europa più unita e più solidale pure sotto il profilo di una rete strutturale che agevoli movimento di persone e di merci. Questa mozione si rivelerà in tutta la sua fondamentale importanza quanto più il Governo saprà, con il supporto del Parlamento, sostenerla nell'ambito della programmazione delle risorse dell'Unione per il periodo 2014‑2020. Tutte queste motivazioni, rilanciate anche sul grande quotidiano del Sud «La Gazzetta del Mezzogiorno»,

questa volontà si levi con una voce robusta e autorevole che mi consente di dichiarare in modo convinto il voto favorevole del Gruppo PdL. È presente in tribuna la Nazionale italiana di calcio universitaria, in ritiro a Roma, in preparazione delle Universiadi che si svolgeranno a Kazan, in Russia.

nasce dall'esigenza di inquadrare le opportunità che la ridefinizione dei corridoi europei apre per il nostro Paese. Il tema è quello delineato dalla nuova programmazione comunitaria per le infrastrutture costituita dalle reti TEN-T. Le questioni, come correttamente riportato nella mozione, sono già state oggetto di ampio ed approfondito esame nella Commissione di merito e in Aula nella scorsa legislatura, sia per la valutazione di congruità dello strumento programmatorio, sia in ragione, soprattutto, di ciò che non era e non è ancora ricompreso in questo e che, invece, auspichiamo quanto prima venga recepito. Provando a riepilogare, la nuova programmazione comunitaria, com'è stato detto, prevede due livelli: la rete globale o periferica, la cosiddetta *comprehensive Net*, rappresentata dalla totalità delle opere necessarie al collegamento di tutti i Paesi comunitari, e la rete centrale o *core Net*, rappresentata essenzialmente da quelle infrastrutture prioritarie che costituiscono la struttura centrale dell'Unione europea. Com'è stato sottolineato, differenti sono le attenzioni che l'Unione europea prevede per questi due ambiti, sia dal punto di vista delle tipologie di finanziamento, sia dal punto di vista delle strategie temporali per la loro realizzazione. Ora, una prima considerazione, in sintonia con l'obiettivo della mozione, consiste nella necessità di introdurre alcuni elementi di riflessione

e in parte esistente dell'Europa, quella centrale, appunto, il cui completamento e ammodernamento è sicuramente un elemento di straordinario rafforzamento dell'Europa già forte, quella cioè rappresentata dalla cosiddetta area della «banana blu», dalla primordiale definizione, ha già conosciuto una tale fortuna da riscontrare, non a caso, il progressivo ampliamento del suo ambito di influenza. Lo stesso corridoio adriatico-baltico e la richiesta dell'istituzione di una nuova macroregione adriatico-ionica nascono, appunto, come naturale evoluzione di espansione di quest'area forte. un'area sicuramente destinata a massimizzare i benefici di ulteriori investimenti, ma che probabilmente - e qui è il punto - non rappresenta al meglio quella che era l'iniziale strategia che l'Unione europea si proponeva, quella cioè di un Continente capace di conciliare sviluppo e coesione sociale, progresso e redistribuzione di reddito, sviluppo equilibrato tra regioni centrali e regioni periferiche e marittime. e regioni periferiche e marittime. Il fatto che le infrastrutture strategiche prioritarie, ricomprese nel corridoio adriatico-baltico, si interrompano a Ravenna palesa l'aspetto che maggiormente contraddice proprio quel principio basilare e costituivo di un'Europa che, da Lisbona in poi, si prefiggeva l'obiettivo di unire se stessa per riequilibrare i differenti livelli di sviluppo e, nella prospettiva, collegare anche i Paesi con essa confinanti. In questo senso l'esclusione dei collegamenti con i Paesi extracomunitari rischia di determinare, oltre che la perdita di una visione strategica che l'Unione europea ha sempre avuto, con lo sviluppo del processo di allargamento iniziato a partire dalla metà degli anni '90 e poi proseguito con maggiore intensità nei primi anni 2000, anche la perdita di una straordinaria occasione di sviluppo. Nella precedente programmazione, infatti, questo principio era rappresentato, com'è stato giustamente ricordato nella mozione Tomaselli, dal corridoio 8 Bari-Varna, che nella nuova programmazione viene invece soppresso. Il corridoio 8 Bari-Varna costituiva un motore propulsivo di esportazione e di redistribuzione di benessere, ma anche un potenziale fattore di pacificazione per l'area mediterranea che, invece, con la nuova strategia di sviluppo delle reti TEN-T, sembra essere messo in discussione. Allora è essenziale che l'infrastrutturazione, in specie quella ferroviaria finalizzata principalmente, com'è stato ricordato, all'alta capacità, non si interrompa a Ravenna ma prosegua per tutta la dorsale adriatica fino a collegare anche le regioni ioniche. La seconda riflessione che voglio porre all'attenzione dell'Aula, anche questa ben impostata nella mozione, prende le mosse dalla filosofia sottesa alla nuova programmazione. Una programmazione delle opere che, come abbiamo visto, rischia di essere, oltre che eccessivamente centralista, anche basata su una più accentuata concentrazione dello sviluppo degli investimenti infrastrutturali rispetto invece alla necessità di una loro più ampia diffusione e redistribuzione. La previsione della trasversale Napoli-Bari, prevista nella nuova programmazione, costituisce in questo senso una grande opportunità di collegamento tra aree a significativa densità abitativa e tra realtà economiche di particolare interesse. Tra l'altro, la previsione della nuova trasversale Bari-Napoli può, anche senza l'ex corridoio 8, farne vivere l'obiettivo di fondo, quello cioè di un collegamento con le regioni dell'altra sponda adriatica, promuovendo così lo sviluppo di nuovi traffici per le regioni periferiche e marittime che conoscono attualmente ancora ingiustificati e ingiustificabili differenziali nei tassi di crescita. Aggiungo, ovviamente, che tutto questo ragionamento che oggi facciamo per la sponda adriatica ha il suo naturale corrispettivo anche per quella tirrenica, a partire dal completamento e dalle realizzazione di altre trasversali altrettanto importanti per lo sviluppo equilibrato e armonico del Paese. Mi riferisco alla Orte-Falconara o alla Grosseto-Fano, o a quella segnalata dall'ordine del giorno a prima firma del senatore Razzi, la Roma-Pescara, che ovviamente condividiamo, e le cui compromissioni o lo stato di degrado fanno del nostro Paese centro-meridionale, se mi si passa questa rappresentazione perfino un po' caricaturale, un Paese voltato di spalle e appoggiato all'Appennino. Collegare a più latitudini la costa tirrenica con quella adriatica, realizzando quello che si definisce «un ponte di terra tra due mari» ricchi di traffici e di relazioni, rappresenta una visione alta dello sviluppo a cui non dovremmo rinunciare, nell'interesse delle potenzialità per il nostro Paese ma anche più in generale nell'interesse dell'Unione europea. Non dovremmo cioè rinunciare alla visione di un collegamento che prolunghi le infrastrutture, infrastrutture che oggi si arrestano invece nella zona centrale del nostro Paese rischiando talvolta di farne «una terra di mezzo» dove si peggiora e si compromette ulteriormente il collegamento tra il Nord e il Sud del Paese, ma soprattutto privando con esso l'Unione europea di una propria vocazione euro-mediterranea. del senatore Tomaselli ha il pregio di richiamare l'attenzione su un'area geografica che ha significative potenzialità di sviluppo e ne tratteggia le giuste priorità. Un mare che è apparentemente chiuso in realtà offre straordinarie occasioni di aperture, tanto in termini di collegamento e continuità per il nostro Paese quanto di relazioni e traffici con i Paesi che vi si affacciano. Collegare tutto ciò che si affaccia su questo mare e unire queste realtà ai principali nodi logistici dei mercati europei costituisce una doppia e reciproca opportunità di sviluppo. Il mar Mediterraneo da tempo ha riscoperto una sua centralità internazionale proprio in ragione della sua attraversabilità dovuta ai traffici che dal *far east* lo solcano nella rotta Suez-Gibilterra, ma anche per le potenzialità di traffici che l'Europa può intrecciare con i nuovi mercati di sviluppo, da quelli mediorientali, a quello balcanico e, in ultimo, ma non meno importante, quello con l'Africa del Nord. Valorizzare queste potenzialità, crederci davvero, vuol dire investirci in termini di relazioni, ma anche materialmente in termini di infrastrutture. Un investimento che non si deve proporre un ritorno solo a breve e medio termine, ma un ritorno più certo in termini di pacificazione di un'area ancora oggi assai tormentata, e soprattutto nella logica di un reciproco maggiore benessere determinato dalla messa in relazione delle reciproche scarsità complementari alle reciproche ricchezze. Collegare l'Europa, costituisce l'obiettivo della nuova programmazione dei corridoi TEN-T. A nostro avviso, ciò significa lavorare per renderla raggiungibile, ma anche lavorare per la costruzione di ponti verso il futuro, verso nuove relazioni, verso nuovi traffici, verso un nuovo sviluppo di pace e di benessere. Per tutti questi motivi votiamo con assoluta convinzione

Senatrici e senatori, secondo quanto già comunicato per le vie brevi ai Gruppi, l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con la votazione a scrutinio segreto di nove senatori effettivi e nove

del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi al Governo affinché si proceda alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per le aree della Lunigiana e Garfagnana, così da permettere la migliore gestione del dopo terremoto. *(Brusìo).*

Dallo scorso venerdì, infatti, quel territorio vive in una condizione di disagio e paura non solo per la scossa principale, ma per lo sciame sismico, che da allora investe un territorio molto vasto, che va dalla Toscana alla Liguria, all'Emilia Romagna. Non vi sono state vittime, anche se la scossa è stata di grado elevato (pari a 5,2 punti della scala Richter) e questo è dovuto in parte anche al lavoro di di prevenzione che si è fatto dopo il terremoto del 1995, da parte dei Comuni, ma anche della Regione. Moltissimi sono, comunque, le case e gli uffici pubblici inagibili o lesionati. La macchina della protezione civile si è messa subito in moto, garantendo un primo aiuto alla popolazione colpita, ma è doveroso che il Governo si impegni da subito

agli ingenti danni, è assolutamente necessario che si proceda allo stanziamento di adeguate risorse in tempi ristretti, per permettere un pronto ritorno alla normalità. È necessario per il futuro dotare di adeguate coperture finanziarie l'attività della protezione civile, affinché possa intervenire prontamente sulle emergenze, con un fondo apposito, senza scaricare con varie accise regionali il relativo

non si può più perdere tempo e non si può rischiare. Il Governo deve dare un segnale importante sottraendo al vincolo del Patto di stabilità dei Comuni i fondi per gli interventi di messa in sicurezza delle scuole e degli edifici pubblici. È fondamentale che in un Paese come il nostro, fortemente esposto al rischio sismico, siano forniti ai cittadini gli strumenti per difendersi e per prevenire le catastrofi, oltre che per garantire tutto l'aiuto necessario una volta che le calamità naturali si siano verificate. Auspico che gli sgravi fiscali per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici contenuti nel decreto-legge ecobonus siano estesi come - richiesto dal Gruppo del Partito Democratico - agli interventi di sicurezza sismica. Mi appello, inoltre, anche agli ordini degli ingegneri e dei geologi affinché mettano oggi a disposizione le loro competenze in questo stato di emergenza, così come è avvenuto in Emilia-Romagna. In conclusione, dobbiamo essere più che mai consapevoli, soprattutto per quanto riguarda questo territorio e in generale per il nostro Paese, di vivere in una condizione di permanente sismicità. Proprio per questo è quanto mai prioritaria e non più procrastinabile l'attivazione di un piano strategico strategico per la messa in sicurezza delle zone a più alto rischio.

coordinatore e direttore scientifico di Neurothon, il quale ha informato che la prima fase della sperimentazione del trapianto di cellule cerebrali in sei pazienti è stata completata senza esiti negativi e senza effetti collaterali. Questo dato ci propone un'informazione di cui dovremmo fare tesoro non soltanto per risultarne oggi orgogliosi, ma per capire, come

sarebbe permesso ad una tecnica messa a punto nel 1996 - quindi ben 17 anni fa - di procedere con maggiore celerità per riuscire a dare una notizia così importante 4-5 e forse più

e che spesso devono ricercare i fondi direttamente da privati o da singoli cittadini, nella condizione di lavorare celermente, con il dovuto rispetto, senza patemi d'animo e con il sostegno vero della pubblica amministrazione italiana, del Governo italiano e di tutto il Parlamento. Investiamo nella ricerca, in queste ricerche, che danno valore alla vita umana e al lavoro di tante persone

Presidente, colleghi, mi scuso se intervengo in merito a un argomento che ha ben poco di politico, ma riguarda la funzionalità dei nostri lavori d'Aula. Da alcuni decenni ho scelto di spostarmi con la bicicletta per tutti i movimenti della giornata, e uso la bicicletta anche per venire in Senato.

Presidenza segnala la questione agli Uffici competenti.

sezione di Sinistra Ecologia e Libertà, del Partito Democratico e della Confederazione generale del lavoro sono stati devastati da un incendio ad opera di ignoti a Roma, nel quartiere Trionfale, in via Pietro Giannone. La nostra città è reduce da una campagna

sarebbero cessati e avremmo potuto considerare un modo e una relazione, anche nel confronto politico, che escludessero assolutamente episodi di questa natura o consimili.

Credo che non solo, come si dice sempre in questi casi, non dobbiamo abbassare la guardia, ma dobbiamo - anche per quello che ci compete - tenerla alta e determinare atti che consentano

nell'ambito del rispetto, non solo formale, delle condizioni democratiche. Invito poi, nelle sedi adeguate, a far sentire il peso unitario di quest'Assemblea per contribuire ad interrompere sul nascere un possibile tentativo di *escalation* da questo punto di vista.*(Applausi

che riguarda un problema gravissimo che vivono alcune realtà nostre, della Sicilia. In particolar modo, faccio riferimento

gli ospiti che ci vivono sono riconosciuti come persone, la considerano una casa famiglia. Essi possono essere aiutati nel recupero, così come prevede la nostra Carta costituzionale, svolgono dei corsi professionali, artigianali

tutto il lavoro straordinario svolto, che è poi quello che andiamo dicendo che vogliamo quando ci preoccupiamo delle carceri sovraffollate, o ci disperiamo per l'ennesimo suicidio di un detenuto (e sappiamo che il sovraffollamento è una causa scatenante),

nella mentalità e nella logica, che io non condivido, del risparmio in questo senso) rischieremo anche delle infrazioni. Infatti, tutto ciò non sarebbe dovuto accadere se si fossero fatti i lavori nel carcere della città contigua di Ragusa; ebbene, quei lavori non sono stati neanche iniziati.

ha già il destino segnato. Noi potremo recuperare quel ragazzo se resterà in quella casa, ma se sarà trasportato e buttato non so dove, quella bambina, Maria Sole, non incontrerà più suo padre o lo vedrà molto raramente, e purtroppo ricalcherà lo stesso percorso. Allora, questa è la prevenzione;

vivere questa meravigliosa avventura, dobbiamo veramente chinare il capo davanti a tutto ciò oppure possiamo gridare alto il nostro desiderio di rispetto della Carta costituzionale, che tutti diciamo di venerare.

a Gragnola e in altre zone, ed è lì - ripeto - che bisogna andare. Occorre dare le risorse non alle amministrazioni ma ai cittadini che, da soli, le recupereranno e riusciranno a rimettere a posto quei borghi

considerazione. Sono sicuro che la procura di Massa non aprirà fascicoli contro la scienza, come è accaduto all'Aquila, non si condannerà chi non ha previsto i terremoti, perché certe sentenze non vanno rispettate, come quella dell'Aquila, dove i più grandi scienziati sono stati accusati di non aver saputo prevenire i terremoti, facendo un danno di immagine all'Italia incommensurabile. Noi ci auguriamo che ci si rimbocchino le maniche e seriamente si cerchi la ricostruzione e chi fa danni, come è accaduto all'Aquila,